che si è verificata circa un paio di ore fa, in occasione dell'elezione del Presidente della Commissione speciale per la In occasione dello scrutinio, si è riscontrato il raggiungimento della maggioranza prevista più un voto in testa al senatore Pianetta, per un totale di 14 voti, mentre il candidato del centro-sinistra ha raccolto 11 voti. Nonostante questo scarto, a causa della presenza anomala di una scheda in più rispetto al numero dei votanti, effetto sicuramente anomalo, ma secondo noi - e ci ci auguriamo anche ad avviso della Presidenza, al cui vaglio è stata posta la vicenda - non influente ai fini della determinazione del *quorum* previsto, non è stata proclamata definitivamente l'elezione del senatore Pianetta.

noi abbiamo ridotto già notevolmente gli emendamenti anche questa mattina e stiamo rispettando i tempi previsti dal contingentamento disposto dalla Presidenza. Abbiamo accettato questo contingentamento che prevede la possibilità di concludere serenamente i lavori nella giornata di domani.

che si possa trattare - perlomeno, così mi sento di dire - di un incidente piuttosto sgradevole. La Presidenza del Senato, comunque - come lei ben sa - è attivata immediatamente per sciogliere questo spiacevole nodo che si è determinato nella Commissione. Confidiamo in una soluzione positiva

di uno spiacevole incidente. Vi è un principio, ormai consolidato nella giurisprudenza, quello della conservazione del risultato utile per tutto ciò che riguarda questioni di carattere elettorale: ritenevamo quindi che il voto espresso dalla Commissione, proprio per come numericamente si era andato determinando, non potesse che essere rispettato. Affronteremo serenamente,

Vorrei segnalarle, signor Presidente, che le votazioni si sono tutte svolte sotto il controllo dei segretari di Commissione, che hanno provveduto alla consegna delle singole schede; quindi nulla può in alcun modo essere imputato ai componenti della Commissione che in quel momento stavano procedendo alla votazione. a maggior ragione, non si può che essere trattato di un evidente incidente di percorso, legato semplicemente alla presenza di una scheda bianca in più. Ripeto che non è dato quindi comprendere per quale ragione si sia ritenuto di adottare una decisione che si discosta significativamente da quanto costantemente è stato affermato in materia.

nella concitata situazione in cui ci troviamo, non guardiamo con serietà. Mi riferisco al conflitto aperto tra la Turchia e la popolazione curda. Sono giorni che si svolge un conflitto in armi, il quale ormai si sta svolgendo con tutta la crudeltà tipica di un conflitto armato. Esso ha già mietuto varie vittime e oggi le agenzie battono notizie gravi di incursioni dell'esercito turco nei territori iracheni dove si trovano i curdi, di scontri con le milizie curde e di ulteriori vittime.

Questo ci dice quanto sia fragile la situazione in quell'area e quanto questo conflitto possa ulteriormente alimentare l'incendio che divampa in Medio Oriente. La preoccupazione riguarda la sottovalutazione con cui guardiamo a questa situazione e anche il modo con

è di tutta evidenza che nell'arco delle prossime venti ore si dovranno votare tutti gli emendamenti. Per evitare qualunque dubbio, ho già chiesto ai colleghi dell'UDC di non procedere ad illustrare gli emendamenti che abbiamo presentato, salvo pochissimi casi in cui vi sono particolari ragioni di politica generale Non vi è, a nostro giudizio, alcun motivo per cui si possa andare al voto di fiducia. Lo dico per evitare che si continui ad affermare qualcosa privo di senso costituzionale.

al CNEL. Essendo stati ristabiliti la verità e il diritto, ringrazio il Presidente per la solerzia con cui ha convocato la Giunta e revoco la mia irrituale autosospensione. Quindi, tornerò a presiedere per venire incontro anche alle richieste del collega D'Onofrio, in modo che i lavori riprendano con una certa celerità e che nessuno possa essere chiamato a porre una fiducia che non ha ragion d'essere

dei pareri espressi nella seduta antimeridiana. Mi riferisco all'emendamento 5.47 che nello stampato risultava a firma Tomassini, Bianconi ed altri; si tratta invece di un emendamento della Commissione e quindi io devo cambiare - lei comprenderà, Presidente - il parere da negativo a favorevole. Per quanto

pensiamo che la ripartizione del 100 per cento a carico della filiera risulti abbastanza inaccettabile, in quanto da una parte abbiamo le imprese farmaceutiche

Ci sembra una specie di esproprio di Stato, qualcosa che ha a che fare con l'abitudine che avete, con i Casarini e quant'altro, agli espropri sociali.

si è presentato un senatore della maggioranza, venendo qui di corsa. Allora, quello che volevo dire è che il voto era stato espresso da me, mi trovavo in prossimità della porta e non ho fatto in tempo a raggiungere di nuovo il mio posto per un problema visibile che ho ad una gamba. Volevo solo dire questo, affinché nessuno potesse immaginare

ha il dovere, in votazioni che avvengono con margini ristrettissimi per definire maggioranza e opposizione, a tutela del Senato e anche di coloro che votano, di far sì che il voto avvenga nella maniera più regolare possibile. Lei ha dato adesso una spiegazione adesso di quanto è avvenuto, ma la Presidenza aveva il dovere di intervenire essendo quella la situazione che è stata descritta da lei stesso.

Del Pennino, sistematicamente appaiono sei voti e non cinque quanti sono i senatori seduti. È dall'inizio che avviene

Senatore Nessa, quella è la scheda del senatore Barba; la prego di estrarla perché il senatore Barba è assente. La richiamo all'ordine, senatore Nessa, non si può permettere di fare cose del genere verso la Presidenza del Senato.

Signor Presidente, intervengo su due emendamenti di identico contenuto che affrontano una questione molto importante e ringrazio i colleghi Monacelli e Polledri per averli portati all'attenzione dell'Assemblea.

prevedeva il blocco biennale dei prezzi dei farmaci. Era il tempo in cui si diceva molto per propaganda, ma in parte anche con verità, che la gente non arrivava all'ultima settimana del mese quando oggi è invece noto che si va in villeggiatura per tutto il mese.

Essi sostengono anche che le aziende farmaceutiche non possono aumentare indiscriminatamente, nel mese di gennaio di ogni anno, questo tipo di offerta al cittadino.

difficile trovare contrarietà. È una norma che non costa al cittadino, anzi, lo fa risparmiare; è una norma che non costa allo Stato; è una norma di giustizia rispetto all'*escalation* dei prezzi. In questo caso ci occupiamo dei farmaci, avremmo voluto occuparci anche di altro, ma il Governo ha deciso di non permettercelo con il cosiddetto

una questione di tale importanza possa sfuggire. Signor Presidente, vorrei che il Ministro facesse un passo in avanti rispetto a questa proposta, consentendo finalmente ai cittadini di sentirsi garantiti, soprattutto di fronte agli aumenti dei prezzi.

*(AN)*. Signor Presidente, poc'anzi mi sono permesso di chiedere la controprova sulla precedente votazione e o non sono stato ascoltato o, ascoltato,

Presidente, per l'immissione in commercio dei generici o farmaci equivalenti ora basta semplicemente un'autocertificazione. Ciò é stato oggetto purtroppo di molte truffe perché basta costituire una società a si verifichi ancora la persistenza del brevetto, qualcuno può immettere illecitamente farmaci sul mercato. Noi riteniamo che questa dichiarazione oggettiva dell'Ufficio italiano brevetti nulla costi, porti più chiarezza e diminuisca le truffe. Non riusciamo a comprendere il perché di un parere negativo del relatore e del Governo e, pertanto, noi voteremo favorevolmente

Entrambi gli emendamenti, sia quello del senatore Tomassini ed altri che quello del senatore Polledri, risultano integrati esattamente dalla stessa frase,

altrimenti, è difficile escludere un emendamento non pertinente alla promessa fatta precedentemente. Vi è, cioè, l'intenzione di favorirlo? Stiamo parlando, cari colleghi, di 5.000 patologie rare,

Sull'eventuale trasformazione in un ordine del giorno - se ho capito bene l'intervento del senatore Massidda - si chiede un'ulteriore specificazione rispetto al quesito posto. Invito, dunque, il relatore e la

del regolamento sulle malattie rare; dall'altro, un impegno nella ricerca sui farmaci orfani.

Presidente, illustrerò brevemente l'emendamento 7.0.500, che fa riferimento al rafforzamento dei collegamenti con le isole minori.

Pensiamo, ad esempio, alla benzina e a cosa si è fatto negli anni scorsi: due Regioni, l'una confinante con la Slovenia, cioè il Friuli, e l'altra confinante con la Svizzera, cioè la Lombardia, hanno potuto dividere il costo degli idrocarburi

queste provvidenze ai Comuni di confine servono anche a temperare quelle disfunzioni e ad evitare che il Parlamento debba, magari ogni mese, pronunciarsi su *referendum* di popolazioni che liberamente decidono di passare da una Regione all'altra.

le isole di Lampedusa e Pantelleria, ma anche di Favignana, oltre che le isole Eolie. Ritengo che questa attenzione nei confronti delle isole minori vi debba essere. Le isole minori non debbono essere frequentate soltanto nel mese di agosto, quando tutto e bello e tutti vanno a fare le vacanze. Bisogna pensare a queste isole anche quando queste devono vivere la loro vita

Credo sia arrivato il momento di risolverlo definitivamente. Quindi, ritengo non vi debba essere divisione tra maggioranza e opposizione di fronte ad un problema del genere, che suscita un malessere profondo in molti Comuni di confine, come ricordava giustamente il collega Divina. Prego pertanto i colleghi della maggioranza di farsi carico in maniera veramente seria del problema, che è particolarmente sentito.

che sostengono questi emendamenti che non è volontà perversa del Governo escludere le città di Torino e di di Palermo e quindi non considerare anche i collegamenti con i piccoli centri, ai quali guardiamo con grande attenzione. È soltanto che il riferimento alle altre grandi città (Milano, Roma e Napoli) è obbligatorio farlo in questo provvedimento, perché, a differenza delle città di Torino e Palermo, non sono incluse nella Legge obiettivo che era stata inserita nella finanziaria precedente.

che rientrano nell'ambito della programmazione prevista dalla Legge obiettivo, i soldi sono già stanziati in finanziaria. Per quanto riguarda, invece, le metropolitane di Roma, Napoli e Milano, si fa fronte con questo decreto e sono soldi finalizzati all'utilizzo nel 2007. Quindi, chiederei al senatore Ghigo di ritirare

Ovviamente è un tema di grande rilevanza, però mi sembra che il decreto già preveda alcuni finanziamenti non irrisori per la realizzazione di tali infrastrutture.

del trasporto pubblico tra Sicilia e Calabria. Al riguardo, però, vorrei segnalare che viene prevista una copertura non idonea, che non può essere utilizzata, perché si prevede di aumentare i risparmi di spesa relativi al contributo dovuto all'Unione Europea. Si tratta di un'operazione che non possiamo fare, perché sono risparmi non decisi dal Governo ma in altra sede.

ci sono Regioni che possono ricevere, ci sono città metropolitane che hanno problematiche e le problematiche degli altri non esistono. Mi sembra assurda la situazione che si sta creando in questo momento sui due emendamenti. Dico no al ritiro, chiedo il voto elettronico e chiedo, se possibile, di fare mio

il 5.0.500, nel quale, al comma 2, si fa riferimento ad un onere di due miliardi di milioni di euro. Non so nemmeno

esse hanno scoperto che lo stanziamento, previsto dal comma 1152 della scorsa finanziaria, era assolutamente scoperto perché il FAS era stato impegnato molto più di quanto fosse la sua consistenza reale e che le destinazioni erano

onde non costringere i senatori tutti, di maggioranza e opposizione, ad impegnarsi nelle proposte di utilizzo dello stesso FAS che, invece, il Governo ha già abbondantemente utilizzato. Evitiamo di prenderci in giro anche tra di noi dal momento che voi avete già preso

Presidente, ho ascoltato l'invito al ritiro rivoltomi dal relatore, ma non posso accoglierlo proprio perché non condivido il merito delle sue argomentazioni. Il relatore ha sostenuto, giustamente, che questi interventi sono relativi alla

Senatore Eufemi, alla sua destra, leggermente in alto, c'è una tessera di un senatore fantasma. Di chi è quella scheda? La può togliere, per favore?

diversi giorni continuativamente è dovuto non solo e non tanto all'inadeguatezza dei mezzi, quanto all'inadeguatezza delle strutture. Il Ministero dell'ambiente continua a respingere le valutazioni di impatto ambientale per la messa in sicurezza dei porti delle isole minori. Se consideriamo cittadini non di serie B ma di serie Z in questo caso gli abitanti delle isole minori, che durante l'inverno devono essere costretti a rimanere tagliati fuori dal resto del contesto nazionale, allora diciamo chiaramente che vogliamo che restino penalizzati in quel modo. Le isole minori, a mio giudizio, hanno cittadini residenti che meritano, al pari di tutti gli altri residenti di questa nazione, di poter essere considerati cittadini con con diritto alla mobilità. Allora, approviamo questo emendamento e interveniamo ulteriormente, per quanto possibile, nei prossimi strumenti legislativi per risolvere questo gravissimo ed annoso problema.

Non so se le colleghe della maggioranza sanno che da molti anni, ad esempio, a Lampedusa non nasce più alcun bambino. Sono anni, anni e anni che a Lampedusa non nascono bambini: come mai? Forse perché i lampedusani non sono capaci più di fare bambini? Fortunatamente no, ma le puerpere, le mamme,

di una terra che è lontanissima dalle nostre plaghe, ma che vive esattamente gli stessi problemi di abbandono da parte dello Stato centralista. Di più, Di più, c'è un costo enorme da parte dei cittadini di Lampedusa per poter andare avanti e indietro rispetto al resto del territorio nazionale; nazionale; oltre a questo danno, vivono la beffa di vedere un'unica categoria di cittadini, anzi non ancora cittadini ma di soggetti che invece vengono trasferiti gratuitamente nel resto del territorio nazionale, che sono i clandestini e gli extracomunitari. Questa è la situazione di quest'isola. Mi rendo conto - mi rivolgo al relatore - che

considerato ammissibile dalla Presidenza, di questo stiamo discutendo, anche se a lei non piace. Allora, all'interno di questa discussione vorrei capire dal relatore se c'è

oppure se il relatore e il Governo si sentono di accogliere una trasformazione in ordine del giorno - sempre ovviamente che il presentatore dell'emendamento sia d'accordo ma che non sia il solito atto di indirizzo di quelli che non si negano a nessuno, che sia veramente un impegno al quale il Governo intende rispondere. Perché vedete,

il rafforzamento dei collegamenti con le isole minori. Questo emendamento rappresenta il momento sostanziale di quell'indicazione programmatica.

Commissione affari sociali della Camera aveva approvato una risoluzione nella quale si chiedeva specificamente, oltre ad un concorso per ostetriche per l'isola di Lampedusa e per le altre isole minori, la predisposizione di un punto di pronto soccorso

È vero anche quello che ha detto il collega Castelli, vale a dire che da molti anni nell'isola di Lampedusa ma non solo in quella, non nascono bambini. Ha fatto bene la collega Valpiana a ricordare che il tema non è soltanto di oggi. Mi verrebbe da chiedere ai colleghi dell'opposizione che hanno governato per cinque anni se è vero che non c'è stata natalità in queste isole negli anni precedenti. Evidentemente la responsabilità

i risparmi di spesa previsti nei confronti della Comunità Europea non li decide il Governo italiano. Sono decisi in altra sede. Senatore Pistorio, la risposta del relatore mi sembra precisa. C'è un'intesa e un accordo per quanto riguarda il merito dell'emendamento che lei ha proposto; è evidente che si rinvia ad un'altra formale copertura per far sì che questo impegno che prendiamo qui in Aula sia mantenuto.

Abbiamo posto un problema in questo decreto: di fronte alla grave crisi delle famiglie, in conseguenza del rialzo dei tassi di interessi che si traduce in più costose rate sui mutui soprattutto per quelli accesi a tasso variabile, anziché sperperare risorse in tanti rivoli, abbiamo presentato una proposta concreta che si traduce in un aiuto vero, in un sostegno reale alle famiglie attraverso l'elevazione della detrazione fiscale e l'aumento dell'importo detraibile,

Presidente, sull'articolo 8 ho presentato diversi emendamenti che hanno come nocciolo fondamentale la questione relativa allo Stretto di Messina, alle modalità del collegamento e alla questione dello scioglimento della società Stretto di Messina. Gli emendamenti, come ha ricordato bene ieri il senatore Lunardi, richiamano la responsabilità di questo Governo su una scelta inaccettabile, improvvida e che costerà carissima non solo alle casse dello Stato, ma al destino delle popolazioni della Sicilia e della Calabria. Questa norma dell'articolo 8, che il Governo ha predisposto nel tentativo di dare una soluzione alternativa al tema del ponte, è la dichiarazione plateale del fallimento di quella scelta. È una norma abborracciata, frammentaria, che tiene insieme interventi diversi che non hanno una *ratio* e che non risolvono il tema di un collegamento stabile e strutturalmente moderno tra la Sicilia e il resto del Paese, che non risolvono il tema della cesura del Corridoio 1 Berlino-Palermo, che era considerato rete strategica transeuropea, e che, ovviamente, ci consegnano ad un destino di emarginazione e di ritardo infrastrutturale. Una politica delle infrastrutture alternativa al Ponte, caro ministro Bianchi, noi non la intravediamo. Non vediamo gli investimenti per garantire comunque l'intermodalità, non vediamo gli investimenti per un attraversamento moderno dello Stretto che consenta in un futuro, per quanto lontano, di avere l'alta capacità e l'alta velocità perché lei sa benissimo che le navi traghetto che oggi collegano le due sponde della Sicilia e della Calabria non sono tecnicamente attrezzate, per esempio, al trasporto degli Eurostar che le Ferrovie dello Stato non hanno il benché minimo interesse ad investire nell'ammodernamento del naviglio quando già perdono ogni anno 100 milioni netti, oltre il contributo per la continuità territoriale che il Governo trasferisce alle Ferrovie dello Stato per il costo passivo dell'attraversamento dello Stretto. Oggi, infatti, non vi è alcuna politica degli investimenti delle Ferrovie dello Stato al di sotto di Napoli perché l'aver risolto in termini negativi il tema del Ponte rende inappetibili gli investimenti nella penisola calabrese e abbandona la Sicilia sul terreno degli investimenti infrastrutturali delle Ferrovie. investimenti infrastrutturali delle Ferrovie. Ci sono disinvestimenti sia sulla linea Palermo-Messina, che per quanto riguarda la Catania-Messina nel tratto Giampilieri-Fiumefreddo già programmato ed oggi desertificato per quanto riguarda i finanziamenti. Ma ancor più grave è la grave è la scelta, totalmente politica e assolutamente da sponsorizzazione di una opzione, che è ideologica e non una scelta razionale di sistema,

viziosamente non un circolo virtuoso ma un circolo vizioso che nasce da una scelta originaria. Sono davvero sconcertato dall'aver ascoltato le dichiarazioni del suo collega Di Pietro, che ha definito un'opera da talebani, equiparabile alla distruzione dei Buddha, avere deciso di sciogliere la società Stretto di Messina, perché si tratta di regalare 500 milioni di euro agli studi di ingegneristica che

il Ministro delle infrastrutture, che ha affermato in pubblico queste cose (tra l'altro si tratta di un personaggio politico che ha fatto del rigore la sua bandiera), ritiene davvero che vi sia uno spreco di risorse pari a 500 milioni di euro, questi avrebbe il dovere di dimettersi da questo Governo per una scelta che lui ha giudicato di tale natura. Ma c'è un'altra soluzione c'è un'altra soluzione per Di Pietro e per chiunque nella maggioranza voglia porre riparo a questa scelta senza avventurarsi, come voi ritenete, nella realizzazione del Ponte, ma non pregiudicando questa scelta

piuttosto che sciogliere la società Stretto di Messina e procedere a strane trasformazioni con modalità del tutto incerte (l'emendamento del relatore è infatti assolutamente impreciso),

questo dazio ad un'ideologia imperante che vede nel ponte sullo Stretto un'opera di regime e dimentica che il ponte sullo Stretto è un'opera che ha attraversato i Governi e le *leadership* ed ha segnato l'impegno di Prodi alla Commissione europea, nonché quello

con la partecipazione delle Regioni interessate e dell'ANAS, mantenendo il *know-how*, le esperienze e le risorse di quella società pronti per essere utilizzati quando un ravvedimento operoso e una capacità di ragionare in termini di prospettiva e di rilancio di quell'area territoriale possano consentire di far scommettere questo Paese su una grande infrastruttura strategica,

di chi sostiene queste ragioni? Un grande Paese e un Governo serio avrebbero accettato la sfida e avrebbero ritenuto che realizzare il ponte in modo trasparente ed efficiente sarebbe stato anche un segnale

innestato un volano che avrebbe potuto davvero consentire, attraverso questa infrastruttura, una nuova occasione di sviluppo. Noi siamo legati a quest'opera. La consideriamo una sorta di manifesto politico di un nuovo modo di intendere lo sviluppo nel Sud e continueremo a batterci per essa. Ma ragionevolmente, prendendo atto di questa vostra inclinazione ideologica, accediamo anche ad ipotesi di mediazione, quale può essere ad esempio una società pubblica che tenga insieme l'ANAS e le Regioni interessate, pur di non perdere il titolo a quest'opera.

Nel contempo, vorrei illustrare l'emendamento 8.701/500, non dissimile da quelli del senatore Pistorio e che si muove nel solco dello stesso ragionamento, con qualche argomentazione di tipo diverso. Quando ho visto l'emendamento 8.701 della Commissione, non l'ho condiviso; non soltanto per le ragioni appena illustrate dal collega Pistorio, ma anche perché secondo me è profondamente sbagliato,

vuol dire dover corrispondere un prezzo che si muove nell'ordine di 500 milioni di euro (non parliamo quindi di poche lire) nei confronti di un contraente depositario di un contratto firmato con una società garantita dallo Stato. Pertanto, se non apponiamo se non apponiamo una copertura finanziaria adeguata a tale emendamento, compiamo un'operazione in totale deroga all'articolo 81 della nostra Costituzione. credo sia molto più ragionevole, anche per altri motivi che mi accingo ad illustrare, procedere più che verso la liquidazione della società Stretto di Messina, verso il trasferimento

Prima di tutto, abbiamo un dovere. Quante volte in politica si sente dire che il nostro dovere è liberare e valorizzare le energie che ci sono nel Paese? Ebbene, il ponte sullo Stretto di Messina, certamente in un ambito limitato, è stato il nostro piccolo laboratorio scientifico e tecnologico, in un'area - quella dell'ingegneria civile - che per tanti anni è stata un settore di punta del nostro Paese e ha raccolto attorno a sé grandissime professionalità, consentendo a tanti professionisti del nostro Paese e a molti professori universitari di cimentarsi su un'opera grandiosa, che per loro è stata anche un sogno professionale, scientifico e tecnologico. Ora la maggioranza di questo Paese vuole soprassedere, perché ritiene che non sia il momento di realizzare l'attraversamento del ponte sullo Stretto; ma un dovere lo abbiamo tutti, quello di valorizzare il lavoro di nostri illustri concittadini che si sono impegnati su questo fronte, non già per un loro vezzo, ma perché lo Stato dal 1971, cioè per 36 anni, aveva deciso di muoversi su quel solco.

Senatore Ripamonti, quando si compiono delle scelte politiche, è assolutamente consentito farlo, ma abbiamo un dovere: quello di minimizzarne l'effetto ai fini della collettività, perché queste risorse sono sottratte a qualcos'altro. Una grande stazione appaltante ha molte possibilità in più di attenuare gli effetti negativi che l'eliminazione della società Stretto di Messina provocherebbe ai danni dello Stato: se, con la liquidazione della società, dovremmo pagare, ad esempio, 500 milioni di euro, probabilmente un'attività negoziale sviluppata all'interno della più grande stazione appaltante del Paese servirebbe ad attenuare un simile effetto, oltre a

Presidente, si snoda sulle dichiarazioni del ministro Di Pietro: pochi giorni fa a Napoli, durante un convegno, il ministro Di Pietro aveva suggerito,

probabilmente per tutte le ragioni che ho appena accennato o per parte di esse. Ancora una volta temo che il ministro Di Pietro non adotti comportamenti parlamentari conseguenti ai suoi annunci:

non è un intervento per dare un contributo alla mia città natale. Il porto di Termini Imerese, per una scelta dell'attuale Governo, è stato inserito all'interno dell'autorità portuale di Palermo,

che la sua presenza in Sicilia non veniva sicuramente riconosciuta dal punto di vista economico e della produttività (realizzare un'automobile in Sicilia

Il beneficio è quello di consentire la messa in sicurezza del porto, in modo tale che gli investimenti

consapevoli anche dell'assunzione di responsabilità del ministro Bianchi nei confronti di tale problema, ritenendo che questa fosse una scelta intelligente. Ritengo che il Parlamento, il Governo, questa maggioranza e il Senato della Repubblica non possano fare a meno (tranne che non si stia qui per

ad un momento di crescita del territorio, visto che gli investimenti proposti non sono così sconvolgenti per le sorti di tale provvedimento. Ecco per quale motivo chiedo con forza che questo emendamento possa trovare l'afflato e il consenso dell'Aula del Senato.

l'emendamento 8.200 interviene su una questione decisamente importante: chiede modifiche alla disciplina delle detrazioni di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi.

il Piano nazionale per la riduzione dei carichi azotati e l'auto-approvvigionamento energetico delle aziende zootecniche, di seguito definito Piano. Ai fini della

mozione approvata dalla Camera dei deputati, di autorizzare il Consiglio dei ministri a dichiarare lo stato di emergenza nelle Regioni Calabria e Sicilia in relazione alle condizioni di attraversamento dello Stretto. La gestione dello stato di emergenza sarebbe a carico del Consiglio dei ministri, di intesa con le Regioni interessate. Vengono previsti per la realizzazione delle opere alcuni finanziamenti importanti: al

appunto, di interventi che possono essere risolti attraverso spostamenti di cifre nei fondi speciali di parte corrente e di parte capitale e poi attraverso un'azione legislativa che possa utilizzare questi soldi.

l'emendamento 8.0.500, esso tratta della questione delle zone franche urbane. È un tema che è già stato affrontato dalla scorsa finanziaria

quindi una richiesta di accantonamento dell'80 per cento degli emendamenti. A questo punto mi chiedo se convenga aprire l'articolo oppure

il meccanismo di comunicazione non ha funzionato, per cui non sono riuscito ad esprimere il mio pensiero, del tutto personale, che non impegna il Gruppo, sulla materia esposta poc'anzi anche da senatori siciliani, i quali partono dal massimo per ottenere il minimo pur sapendo che, da questo Governo, né il massimo né il minimo sarà possibile ottenere. Vorrei ricordare a diversi senatori siciliani che il siciliano non è abituato alle questue, neanche quando è indigente, neanche quando è indigente, e contentarsi di modesti ordini del giorno che sappiamo tutti sono carta straccia, non contano niente come le promesse di fare in finanziaria, è veramente riduttivo se non addirittura umiliante. Quindi, la mia personale posizione, anche se dovessimo sfiorare

La mia personale posizione è un invito, ai proponenti dei vari emendamenti e dell'ordine del giorno, a ritirarli tutti perché questo Governo antisiciliano, ma soprattutto antinfrastrutture, è pronto a fare regali a coloro i quali sono pronti a rimodernare e

la proposta di accantonamento dell'emendamento 8.701, approvato in Commissione, sulla questione della società Stretto di Messina spa e, conseguentemente, la proposta di accantonare tutti i subemendamenti

relativa alle conseguenze negative derivanti, appunto, dallo svuotamento del finanziamento per la realizzazione delle opere per il Ponte sullo Stretto di Messina. di Messina. Con questo emendamento della Commissione votato a maggioranza, si propone addirittura la messa in liquidazione di una società che ha commesso in appalto ad un gruppo di aziende, alcune italiane alcune straniere, la realizzazione di quest'opera: società rischia di pagare una penale non indifferente proprio per la mancata realizzazione dell'oggetto dell'appalto. Adesso, addirittura, attraverso la messa in liquidazione, rischia di vedersi sottrarre all'appaltatore che ha vinto quella gara il proprio contraente, il proprio committente. Credo allora che vada fatta chiarezza su tale

Avete svuotato il finanziamento relativo alla realizzazione di questa opera strategica. Adesso in Commissione avete addirittura proposto l'azzeramento del committente, colui che ha stipulato un regolare contratto di diritto privato nei confronti di un appaltatore assumendo obbligazioni di carattere civile. ritengo allora che su questa scelta vada fatta chiarezza non soltanto legislativa, signor Presidente, ma anche politica. Noi desideriamo che il Governo e la maggioranza non sfuggano da questa responsabilità, se l'assumano con un voto trasparente in Aula in questo momento.

Colleghi, c'è un articolo della Costituzione che recita che ciascun parlamentare esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Ogni tanto ci sono interventi che sembrano eccessivamente

ritengo di accogliere l'invito e ritiro gli emendamenti, ritenendo anche che il Governo, sulla materia delle zone franche urbane, saprà fare molto meglio rispetto a quanto fatto l'anno scorso in modo tecnicamente maldestro ed insufficiente dal punto di vista politico.

Prego,

la Commissione prevede che tale contributo non possa comunque superare il costo complessivo sostenuto dal soggetto nell'anno precedente relativamente

moralizzare il settore dell'editoria e dei relativi contributi avrebbe dovuto agire in maniera completamente diversa. Non si doveva sopprimere, come si cerca di fare, attraverso

di non considerare i costi che sono relativi alla produzione e alla distribuzione eccetera. Cosa succede, Presidente? Questa è la nostra osservazione: sottraendo questa parte, la base la base che assume la prerogativa di poter ricevere le provvidenze aumenta di troppo. Tenuto conto, comunque, che c'è un limite che non può essere superato e che è il totale dei costi sostenuti da parte dell'impresa

al giudizio dell'Aula quella parte dispositiva che va da «tale contributo» a «collaboratori». Questo potrebbe essere migliorativo rispetto alle garanzie di spesa, non allargherebbe la base dei percettori e, quindi, sarebbe di migliore garanzia rispetto ai

consente, secondo me, l'introduzione di un sistema migliore per garantire una più proficua utilizzazione delle risorse disponibili a favore dell'editoria.

Nell'annunciare il voto favorevole all'emendamento 10.700/500 e nell'esprimere anche un'opinione favorevole relativamente all'emendamento successivo del relatore, desidero chiarire ai colleghi senatori che, in realtà, dei soldi dei contribuenti una piccola parte finisce a sostegno di queste iniziative editoriali della politica, una parte enorme e gigantesca finisce ad iniziative editoriali che, in qualche caso, sono quotate in borsa e distribuiscono dividendi. Una parte consistente dei dividendi distribuiti a quegli azionisti provengono direttamente dalla tasche dei contribuenti italiani. Questo è l'argomento che stiamo affrontando con questi tipi di emendamento. Signor Presidente, non è un tecnicismo fermarsi a definire una riduzione che, invece, del 7 per cento cento, inserendo un tetto che, in una prima stesura, era riferito soltanto al costo del lavoro, in un settore in cui l'incidenza maggiore viene a determinarsi dal costo di produzione, dalla carta e dal costo di distribuzione. Era quasi un eufemismo mettere un tetto riferito al costo del lavoro perché significava sostanzialmente distruggere quel tipo di iniziativa La correzione che propone il relatore ci trova d'accordo come soluzione di minimo perché almeno riferisce il tetto massimo al costo complessivo di produzione e distribuzione e costo del lavoro. Resta intonso il problema politico del perché si va a piluccare una serie di finanziamenti relativamente modesti a questo tipo di iniziative di editoria, che può essere un po' il sale della politica, c'è il silenzio più assoluto sulle centinaia di milioni che, attraverso le agevolazioni tariffarie e postali, arrivano forma di dividendi ad azionisti privati e che sono pagati con le tasse dei contribuenti. Un'ultima annotazione, signor Presidente. Tra i vari trucchi che emergono spesso ce n'è uno molto banale. era cioè deciso di dare un contributo diretto di trasferimento all'azienda Poste Spa. Ora, per far tornare il *deficit* pubblico quest'anno al 2,4 per cento, come il Governo ha indicato, ed evitare che arrivasse al 2,5 per cento (uno 0,1 di differenza che pare stia molto a cuore alle vestali della contabilità pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre non stanno loro a cuore le decine di miliardi che nascondono nei cassetti), il trucco qual è, signor Presidente? Quello di trasformare il trasferimento diretto alle Poste Spa in un aumento di capitale, in modo tale che tecnicamente, dal punto di vista contabile, va sotto la linea, poiché se è nella forma di aumento di capitale i soldi lo Stato li passa alle Poste, ma formalmente lo Stato ha una partecipazione azionaria. Mero trucco contabile per limare addirittura dello 0,1 per cento il*deficit,* quest'anno, in rapporto al PIL ed evitare una ennesima figuraccia al Governo che ha appena detto che sarà del 2,4 per cento, cioè doppio rispetto a quello che gli andamenti tendenziali,

Questo è il clima nel quale Governo e maggioranza stanno conducendo i lavori dell'Aula, con un rispetto delle istituzioni francamente, a mio parere, molto modesto. Ma ciò che è più grave è che dobbiamo discutere e mediare questa soluzione che condividiamo e che è proposta dal relatore nell'emendamento successivo, mentre non discutiamo delle centinaia di milioni che passano direttamente dalle tasche di lavoratori che pagano le tasse e quando ricevono 1.000 euro al mese netti di stipendio hanno pagato 1.000 euro al mese tra trasse e contributi sociali per andarli a mettere nei bilanci di società quotate che distribuiscono dividendi.

Presidente, onorevoli colleghi, quello che stiamo discutendo è uno degli articoli più interessanti, più importanti di questo decreto‑legge ed è stato riformulato

Il primo rilievo è politico, collega Ripamonti. Se il Consiglio dei Ministri ha approvato la nuova disciplina dell'editoria con la relativa delega al Governo

La seconda valutazione, invece, è specifica. L'UDC ritiene che i contributi all'editoria vadano ridotti e rivisti. Con l'emendamento 10.700 si riduce dal 7 al 2 per cento il prelievo dei contributi diretti di cui al comma 1 il minore gettito è compensato dall'aumento dal 7 al 12 per cento dei contributi indiretti del comma 5. Va osservato però che tale compensazione non funziona, collega Ripamonti, perché riguarda aziende editoriali che chiuderanno proprio a causa della riformulazione del relatore di maggioranza. Da studi letti e da esperienza diretta, il costo per il personale è pari al 25 per cento del costo complessivo; se i contributi non possono superare il costo per il personale dell'anno precedente,

Ma chiuderanno anche, soprattutto, molti giornali di provincia, eliminando un sano e democratico pluralismo dell'informazione che dovrebbe essere tutelato dal Parlamento, se questo intende ancora tutelare la vera libertà di stampa.

che recita: «La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica». Finora questa trasparenza non c'è stata, sebbene l'avessimo chiesta da tempo. Ci voleva un libro recentemente uscito, «La casta dei giornali», per farci capire quanto poco trasparenti fossero i finanziamenti e i contributi ad alcune società editrici. Se proprio volete compiere un'operazione di equità, dimezziamo i contributi indiretti previsti dal comma 5, che invece, amici della sinistra, non avete voluto toccare. Colleghi comunisti della comunisti della sinistra antagonista, colleghi che avete sfilato sabato scorso con i precari e i disoccupati,

della sinistra antagonista, dare 19 milioni al giornale della Confindustria? È giusto dare 10 milioni al quotidiano della FIAT? È giusto dare 19 milioni per sconto di spese postali all'azienda editoriale di Berlusconi? E si potrebbe seguitare. Un milione di persone avete gabbato ancora una volta, e non solo in Commissione; lo state facendo anche in quest'Aula. Non avete, cari amici della sinistra, il coraggio e la forza di alzare la testa, piegati come siete alle logiche di schieramento, senza saper realizzare quell'equità, quella trasparenza e quella giustizia cui l'Italia guarda e che da voi si aspetta, prima ancora che da noi.

condizione nell'intervenire in questa parte del nostro dibattito. Mi trovo, infatti, ad essere d'accordo con alcune delle valutazioni del collega Baldassarri, che adesso vorrei riprendere, soprattutto in relazione alla formulazione dell'emendamento 10.700 della Commissione, e mi

qualche elemento di merito nell'argomentare la sua posizione. È indubbio che stiamo trattando una questione assai complessa. assai complessa. Non potendo sviscerarla totalmente in un contesto in cui si interviene con un emendamento e con una diminuzione parziale delle provvidenze che vanno all'editoria, del tutto evidente che la nostra discussione lascia molto spazio alle interpretazioni, a volte anche eccessivamente estensive, come quella del collega Ciccanti. Il collega Ciccanti saprà certamente che lo Stato spende nel nostro Paese una cifra che va da 700 milioni a un miliardo di euro per l'editoria e che questa spesa si è progressivamente calcificata sulla base di una scelta politica che il Parlamento ha operato, ma che è assolutamente inattuale e anacronistica. Infatti, certe scelte si sono compiute allorquando si trattava di garantire il pluralismo dell'informazione e dell'editoria, di garantire voce alle forze politiche più diverse nel nostro Paese, di assicurare agibilità a quei giornali che non godevano e non godono di una mole consistente di pubblicità e, quindi, tutelare il libero dispiegamento del confronto democratico nel nostro Paese.

dovrà misurarsi con la necessità di una revisione organica degli interventi per l'editoria, perché i grandi sprechi, caro collega Ciccanti, sono sì a monte, dal «Corriere della Sera», «Il Sole 24 ORE» e «la Repubblica» da soli assommano contributi di 60 milioni di euro, cioè l'intera somma che lo Stato spende per i contributi ai giornali politici, ma le provvidenze sono anche

si fa riferimento ad un inasprimento delle somme da decurtare per le spese di spedizione, si fa riferimento esattamente a quella parte di contributi che tanti giornali - ormai di partito assommano, predicando in questo nostro Paese, con un eccesso di disinvoltura, il liberismo politico. Ma si può essere liberali e liberisti quando si prendono dallo Stato 19 milioni di euro, come fa

convergere almeno su un punto; sulla necessità di richiamare il Governo ad un intervento organico e serio che possa essere esaminato con urgenza dal Parlamento, affinché, in un momento in cui si parla di caste, a proposito e molto spesso a sproposito, si possa intervenire anche sul settore dell'editoria. Si tratta di un intervento di moralizzazione

All'ultimo comma di questo stesso articolo 10 era previsto invece un taglio, sempre del 7 per cento, per quelli che in gergo vengono chiamati contributi indiretti a tutte le società editoriali, sostanzialmente il contributo per le spedizioni postali che viene dato dallo Stato a Poste italiane per realizzare tale servizio verso le società dell'editoria. Ora, signor Presidente, tutto ciò avviene sulla base di una legge che è in vigore nel nostro Paese da circa vent'anni questo fondo ogni anno, quale che sia il Governo che in quel momento sta dirigendo la cosa pubblica in Italia, viene sistematicamente, direi inesorabilmente aumentato. Per la verità, anche rispetto alla finanziaria - non disperino - ho l'impressione che l'aumento ci sarà anche quest'anno, ma spero di sbagliare; tuttavia, nel testo del decreto era previsto Ora, ho sentito accorati interventi da parte degli uni e degli altri a proposito del fatto che, certo, un conto è aiutare l'editoria politica, un conto aiutare l'editoria minore, conto aiutare le associazioni *no profit*, che editano pubblicazioni da mandare alle famiglie per sollecitare sottoscrizioni, e così via. Sono tutte attività di grandissimo peso, ma si dice

un contributo che costituisce una parte enorme dei dividendi che tali società editoriali distribuiscono ai proprietari delle stesse stesse e da parte di tutti si sostiene che bisognerebbe intervenire con un'operazione di moralizzazione. Per la verità, signor Presidente, partendo da questa base,

sulla base di una proposta del senatore Montalbano presentata in Commissione, la Commissione, ha pensato però che, fatta questa operazione per i contributi diretti sul comma 1, fosse necessario aggiungere una norma di moralizzazione. La cosa incredibile, Presidente, è che l'abbiamo messa:

della Commissione dice che il contributo non può essere superiore alla somma dei costi del lavoro di grafici, poligrafici, direttori, redattori, collaboratori del giornale che viene editato.

Sul versante della contribuzione indiretta, che è la polpa della spesa pubblica in questo campo, cioè le spese per spedizione postale che si riferiscono anche alle grandi società editrici verso le quali si è menato scandalo negli interventi in questo campo, cosa fa la Commissione rispetto al testo del Governo? Dice il taglio sulle società che hanno un contributo inferiore ad un milione resta al 7 per cento, mentre il taglio sulle società che hanno un contributo indiretto superiore al milione - ce ne sono cinque in Italia, colleghi, e sono quelle che avete nominato voi - diventa del 12. Allora, Presidente, colleghi, adesso Governo e Parlamento faranno la riforma e verrà introdotta una moralizzazione, ma sostenere che il lavoro svolto in Commissione rispetto al testo del Governo non è una accentuazione del processo di moralizzazione e una riduzione di costi significativa per vantaggi che andavano a società che sembrano non averne bisogno, visto che distribuiscono dividendi a go go ai loro proprietari, non è vero. Mi spiace se vi ho fatto perdere tempo, ma credo si dovesse dire la verità

Presidente, penso che una moralizzazione sia necessaria, anche se tardiva, perché in questo Paese ci sono cinque testate che rappresentano precisi interessi dell'oligarchia, anche bancaria e finanziaria, e che lucrano 60 milioni di euro l'anno. La cosa grottesca è che queste cinque testate, periodicamente, svolgono una campagna di mobilitazione dell'opinione pubblica contro le testate di nicchia e contro i giornali di partito, sempre in nome di una presunta moralizzazione. Penso che in questo momento sia quanto mai necessario limitare i contributi indiretti, che, in realtà, sono forme di finanziamento improprio a testate che distribuisco copiosi dividendi ai loro soci.

senatore Carrara,

in dichiarazione di voto sull'emendamento 10.700/500 da me e dagli altri colleghi, e in ultimo, prima della dichiarazione in dissenso del senatore Novi, autorevolmente dal presidente Morando, Italia è contrario all'approvazione dell'emendamento del relatore perché era stato un fatto un buon lavoro in Commissione. Quindi, senza l'approvazione dell'emendamento 10.700/501 rimarrebbe la proposta della Commissione, cioè l'emendamento 10.700, che è certamente migliore di tutto quel che potrebbe nascere con l'approvazione dell'emendamento del relatore che noi volevamo correggere. Non potendolo modificare, a questo punto, meglio bocciare l'emendamento del relatore e ritornare all'ottimo lavoro che avevamo svolto in Commissione con la proposta della Commissione stessa. Non è un'inversione dialettica, Presidente, è una proposta chiara che ha una ragionevolezza credo. *(AN)*. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale sull'emendamento 10.700/501, del relatore che ci pare ristabilisca, come ha già ricordato il Presidente della Commissione bilancio, un equilibrio che altrimenti avrebbe finito, permanendo la precedente formulazione, per venir meno proprio per i poteri deboli dell'editoria, perché questo sarebbe accaduto. A parte la circostanza, per lo meno suggestiva, data dalla comparazione dei costi, che ricordava anche il senatore Ciccanti, tra i costi riferibili ai salari e quelli riferibili alle altre voci che compongono altre spese dell'editoria, sarebbe stato davvero mortificante e irrealistico mantenere la precedente formulazione. Per tutte queste ragioni, Alleanza Nazionale annuncia il proprio voto favorevole.

Dichiaro aperta la votazione.

a quei giornali e a quei periodici che hanno un Gruppo parlamentare presente in Parlamento; *ergo*, si procede a quella moralizzazione da lei

Dichiaro aperta la votazione.

tutta l'Italia ha seguito, ieri sera in televisione e oggi sui giornali, una dichiarazione autorevolissima

«Positive le parole di Bertinotti, chiarito l'equivoco». Sembrava quindi che tra il Presidente della Camera e Palazzo Chigi ci fosse stato il chiarimento politico che in qualche modo tranquillizzava gli italiani.

di fronte a queste dichiarazioni di un autorevolissimo esponente della politica e delle istituzioni, e di fronte ad un falso di Palazzo Chigi che dichiara che è chiarito l'equivoco

Signor Presidente, colleghi, questo è l'ultimo di una serie di emendamenti che andavano tutti nella stessa direzione. Qui avete parlato più volte di moralizzazione. Io non ci credo. Voi non moralizzate proprio niente. Questo è il sistema di moralizzare? Sapete quanti contributi vengono erogati a gente che si presenta con testate fatiscenti: le hanno citate prima

agli organi di partito che hanno la rappresentanza di un Gruppo parlamentare, non di un singolo senatore o di un singolo parlamentare. Questo è quanto vi chiediamo di votare. Naturalmente, vi nascondete, fate come gli struzzi dentro la sabbia, ripeto, poiché siete ricattati.

una continua critica verso i nostri emolumenti: molti direttori di giornale sostenevano che noi guadagniamo troppo. Probabilmente è vero la Lega ha presentato una serie di emendamenti, sia in questo provvedimento che in finanziaria, che mirano a ridurre i costi della politica, ma io credo che dobbiamo moralizzare tutto il settore che gode di contributi pubblici. Questo emendamento prevede

direttori moralizzatori verso la politica che però non moralizzano se stessi. Con questo emendamento prevediamo che i contributi pubblici possano essere erogati soltanto a quei giornali che al loro interno abbiano erogati degli stipendi al massimo pari agli emolumenti dei parlamentari. Credo sia una misura di moralizzazione che il Parlamento dovrebbe condividere: non costa nulla allo Stato, anzi permetterebbe dei risparmi, francamente non ho capito bene per quale motivo

francese, ladina, slovena e tedesca, cioè in tutte queste lingue. Se si sostituisce la "e" con la "o" vuol dire che francese, ladino e sloveno valgono tanto quanto la sola lingua tedesca.

e per oltre la metà del tempo di trasmissione, programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca. Quella "e" è messa semplicemente alla fine di un'elencazione, che per il resto ha la virgola. Se ci mettiamo una "o" non cambia la sostanza, purché ci siano

Signor Presidente, a quest'ora corriamo il rischio di scrivere cose che non corrispondono alla nostra volontà. Se ho ben capito, le preoccupazioni del senatore Peterlini non sono quelle che apparivano fino a questo momento e rispetto alle quali il Presidente della Commissione bilancio aveva detto essere del tutto indifferente sia la "e" che la

perché quella «o» è in alternativa alle altre lingue. La cosa è talmente palese che è inutile che cerchiamo di girare intorno al problema: cambia l'emendamento. Tra l'altro, con tutto il rispetto nei confronti del collega Peterlini,

Signor Presidente, il buon senso mi spinge a sostenere le tesi del senatore Peterlini che non mi sembrano così campanilistiche, ma ispirate a criteri di giusta tutela di minoranze linguistiche. Bisogna, perché questo testo, senatore Peterlini, è scritto con i piedi e, dopo questa discussione, si presta ancora di più ad essere contestato nell'aula di qualunque tribunale perché grammaticalmente

La seconda lettura, egualmente possibile dal punto di vista della grammatica italiana, è che bisogna trasmettere in tutte queste lingue; infine, la terza lettura, che è quella che credo abbia attratto per prima l'attenzione del senatore Peterlini, è che, mentre è possibile trasmettere o in francese o in ladino, bisogna, invece, trasmettere in sloveno e tedesco. Ciò è assurdo perché la finalità è quella di garantire minoranze che, in questo caso, non si

non mi avessero detto che non è più possibile. Io consiglierei di ritirare l'emendamento e di riformularlo alla Camera, assicurando anche la massima comprensione. Altrimenti, questo in tribunale porterà a un mare di contestazioni.

Presidente, volevo solo fare una proposta che, secondo me, risolve il problema attraverso un piccolo aggiustamento del testo. La «e» rimane tale, quindi, non cambia in